"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Presidente, azzardo e autovelox sono solo due diversi modi di succhiare soldi agli italiani. Sia chiaro che il Movimento 5 Stelle chiede e vuole sicurezza sulle strade, ma qui c'è qualcosa non torna: l'autovelox, il rilevatori semaforici vengono introdotti con la specifica ed espressa finalità di aumentare la sicurezza e possono essere installati solo a determinate condizioni. Inoltre, i proventi delle multe raccolte devono essere destinati alla sicurezza. Qui qualcosa però non torna: se un autovelox è piazzato in modo visibile e segnalato, gli automobilisti rallentano e la sicurezza aumenta. Se viene posto in maniera diversa, le multe aumentano e la gente muore, perché qualcuno ha sacrificato la sicurezza al fare cassa. Analogo discorso vale per i semafori: come dice la letteratura internazionale si pone un tempo di giallo di otto o nove secondi, si ha il maggiore effetto preventivo; ma, se lo si riduce a tre secondi, aumentano le multe e si sacrifica la riduzione di incidenti, lesioni e morti. Questa non è prevenzione: è predazione. Con questa manovrina abbiamo un altro indicatore del fatto che il Governo deroga dalle finalità dichiarate e riconosce e ammette spudoratamente che siffatti apparecchi non sono introdotti per la salute e la sicurezza dei cittadini, ma per fare cassa e consentire agli enti locali di fare cassa a fronte dei tagli che il Governo impone a livello locale. Una manina ha infatti introdotto un articolo un articolo aggiuntivo che prevede che gli enti locali possano destinare a fini diversi le somme raccolte, provenienti dalle multe.

e non ad altri scopi. Con questo intervento sono liberi tutti: i Comuni potranno fare cassa meglio e di più e mettere le mani nelle tasche dei cittadini, che si vedranno sottratti denari, senza una ricaduta sulla loro sicurezza sulle strade. Su questa vicenda ho chiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di aprire un tavolo tecnico per confrontarci, perché non è chiara nemmeno l'omologazione di questi apparecchi: ci sono delle cose che non tornano e non è chiaro il loro utilizzo. A fronte dell'emendamento, dei deputati, dobbiamo pensare che non c'è la volontà di confrontarsi, perché questo è l'andazzo che si vuol mantenere. Vengo poi alla questione dell'azzardo:

in calo di gettito, perché sopravanzati da "macchinette mangiasoldi" di nuova generazione, ovvero le *videolottery*

Ciò significa che si va a tagliare qualche ramo secco di un settore che già subisce una concorrenza. E dove si va a incidere? Si incide prima dove ce ne sono troppe, dove ce ne sono di più e dove hanno uno scarso rendimento.

svincola i concessionari delle sale bingo dal rispettare l'obbligo di mantenere costante la sede in cui operano, come previsto nelle convenzioni di concessione. esistenti in Italia, questo provvedimento andrà a toccare un'unica sala in Romagna. Non risulta che suddetta sala debba avere un trattamento privilegiato rispetto agli imprenditori. imprenditori. Se sopraggiungono fatti di causa maggiore, un imprenditore si adegua o chiude. La sussistenza di una concessione non può garantire un privilegio, laddove essa prevede degli obblighi. Qui si stanno togliendo degli obblighi mantenendo i privilegi: non è più rischio d'impresa, è protezionismo di Stato. colleghi, la cosiddetta manovrina riveste una particolare importanza nell'attuale fase congiunturale in quanto, oltre ad assicurare il controllo dei conti pubblici, promuove, attraverso un articolato insieme di misure, interventi per accompagnare la crescita dell'economia e dell'occupazione. Sono numerosi gli interventi previsti, così come è stato sottolineato dal relatore Giorgio Santini, che ringrazio, e da numerosi colleghi. Voglio soltanto segnalare, quali fatti importanti e che determineranno conseguenze assai positive, la parziale disattivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia, le misure per il sostegno alle zone colpite dai recenti eventi sismici del Centro Italia e quelle che affrontano taluni problematiche degli enti territoriali. Il provvedimento può suddividersi in sei aree di intervento: la parziale disattivazione delle clausole di salvaguardia; le misure per il controllo dei conti pubblici; le misure per la crescita; le misure per gli enti territoriali; le misure per il terremoto di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; infine, le misure per l'istruzione e la cultura. Scelgo di soffermarmi sulle misure per il terremoto in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche perché nel dibattito che ha preceduto questo intervento sono state fatte affermazioni assolutamente non congrue. La prima affermazione riguarda la possibilità di intervenire una volta per tutte sui terremoti, così come ha dichiarato qualche collega.

del terremoto del 2009 - ancora oggi, dopo otto anni, abbiamo necessità di legiferare e non perché non solo perché non si è sempre ben legiferato, ma anche perché sorgono esigenze cui di volta

si sta tentando, appunto, di fare questo. Esso, infatti, contiene misure assai significative come - ad esempio - lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge. Vi è poi l'istituzione di un fondo per accelerare le attività di ricostruzione con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687 milioni di euro per il 2018 e 699 milioni di euro per per il 2019, da utilizzare per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni colpiti dal sisma e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1. Inoltre, voglio sottolineare, essendo la prima volta, che finalmente si interviene

Finalmente è stato fatto e bisogna dare atto al Governo e a questa maggioranza di procedere con decisione su materie delicate. Inoltre, sono previsti interventi, ulteriormente ampliati alla Camera, quali l'assegnazione di spazi finanziari volti ad agevolare l'effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione proprio da parte di quegli enti locali colpiti che,

Inoltre, ci sono misure di rilievo tra le quali l'incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e di 132 milioni di euro per il 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite il 24 agosto 2016, anche per consentire l'intervento urgente per la ricostruzione pubblica e privata in quelle aree. Particolarmente importanti sono anche le disposizioni di proroga di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, ed è prorogato dal 16 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 - quindi di più di un anno - il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati. versati. Di particolare rilievo sono anche le disposizioni riguardanti l'istituzione e la disciplina di una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici

carico dei datori di lavoro. La fruizione di queste agevolazioni da parte delle imprese è possibile entro un limite di risorse abbastanza importante per iniziare: si comincia con 194 milioni di euro

per le aree colpite dal terremoto del 2009. In particolare, finalmente si equiparano le funzioni e il trattamento accessorio e salariale degli uffici speciali

con il sostegno del Governo, riusciremo a intervenire nei passaggi successivi e con altri provvedimenti.

questa ulteriore manovra, che vale 3,4 miliardi di euro, rappresenta semplicemente la toppa a un errore di programmazione delle risorse e al buco dello 0,2 per cento del *deficit* generato anche per finanziare le marchette pre-*referendum* che - vi ricordo - avete perso. è così vero che siamo di fronte a un provvedimento che, pur essendo nato per dare un po' di ossigeno agli enti locali, almeno a giudicare dal titolo, rappresenta invece solo un guazzabuglio di proposte assolutamente disorganiche e frutto esclusivamente di un compromesso tra le varie componenti di un Governo francamente stanco,

nuovi buchi, ed è l'ennesimo capitolo di una politica economica che non fa altro che avvitarsi nel circolo vizioso di tagli alla spesa e maggiore burocrazia.

deputata del Partito Democratico è intervenuta inserendo una norma che abroga un vecchio regio decreto del 1931. Per carità, un regio decreto può sempre essere toccato, modificato e corretto, ma in questo caso viene semplicemente abrogato e si crea così un enorme *vulnus* normativo, che sarà riempito con un altro meraviglioso *jobs act* che ogni società di trasporti sottoscriverà per superare l'assenza di norme. Lascerete ancora una volta i lavoratori suddivisi a seconda della loro società di appartenenza.

Noi abbiamo provato a presentare un emendamento per sopprimere questa norma, ma - come ho già detto - questa norma è stata inserita da un'esponente del Partito Democratico che sembra abbia interesse al trasporto privato. Al Senato ci viene detto, da alcuni esponenti, che la norma è comunque una schifezza, ma al Senato verrà posta la fiducia e tutti quanti saranno d'accordo nel farla passare. Questa è una grande prova di coerenza verso il proprio modo di pensare, ma di totale incoerenza nei confronti dei lavoratori. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è interessante che si possano utilizzare noleggi di autobus sempre che siano meno vecchi di dodici anni e si parla di rinnovare il parco mezzi, e va molto bene; si parla di poter assumere controllori per fare le verifiche sui pullman, e va bene; ma non si precisa se sono in carenza di organico, e quindi esternalizziamo e andiamo avanti. riguarda i concessionari autostradali, c'è un'altra marchetta: sull'autostrada A24-A25 si prevede che i contributi che devono essere pagati dallo Stato per gli adeguamenti antisismici possono essere fatti tra dodici anni.

contribuzione nei suoi confronti e la troviamo all'interno di questa manovra. C'è una parte che riguarda i servizi ausiliari del personale ATA, che andava comunque ancora una volta protratta, e su quel versante bisogna andare oltre le misure emergenziali. Tra le misure

Grazie

Vorrei ricordare al Governo che il desiderio di sopprimere questa Camera attraverso il *referendum* costituzionale è stato bocciato dagli elettori italiani. Credo quindi che le alte cariche dello Stato dovrebbero garantire il rispetto delle regole,

Questo provvedimento si è reso necessario perché l'Unione europea ha chiesto al Governo una manovra pari allo 0,2 per cento del PIL (3,2 miliardi) per

di 2.260 miliardi. Tornando indietro con la memoria, quando i Governi del Partito Democratico si sono insediati in questo Paese, il debito pubblico era di 1.905 miliardi; ora siamo a 355 miliardi sopra il il debito pubblico è cresciuto è cresciuto di 43 miliardi. Credo che sia ormai una situazione davvero insostenibile. Tutto questo squilibra il rapporto debito pubblico e PIL perché purtroppo, contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi europei, la crescita resta modesta e siamo a sette punti sotto i livelli pre-crisi, cosa confermata anche dalla flessione del reddito *pro capite* dei cittadini italiani, che a oggi è inferiore del 7,1 2008. Drammatica è anche la situazione dell'occupazione: mentre altri Paesi hanno superato i livelli di occupazione dell'anno 2008, in Italia siamo ad oltre 300.000 unità in meno. La cosa più interessante del provvedimento è che mette nero su bianco una triste verità: dal 1° gennaio 2018 aumenterà l'IVA. Non entro nelle articolazioni dell'IVA da qui ai prossimi tre anni perché solo una mente perversa

l'aliquota agevolata passerà dal 10 all'11,5 per cento e quella ordinaria dal 22 al 25 per cento. Si tratta di 15 miliardi da coprire; non so come questo Paese potrà farlo nei prossimi mesi. questa manovra per 3,1 miliardi di euro è realizzata al 90 per cento sul fronte delle entrate: circa 2,9 miliardi è la differenza tra maggiori entrate e minori spese. La norma che più grida vendetta è quella dello *split* *payment*, con la quale rastrellate circa 4 4 miliardi di euro. I professionisti che forniscono la pubblica amministrazione per tre anni dovranno fare banca allo Stato perché quando vanno a credito IVA non potranno recuperarla. Vi inventate anche un'altra cosa: riducete la possibilità di compensazione dei crediti con lo Stato da 15.000 a 5.000 euro. Già 15.000 euro erano una miseria e voi portate ora la cifra addirittura a 5.000 euro. Siete straordinari perché la "vendete" contemporaneamente

dicendo che sono ridicole anche le norme per il terremoto. Voi sapete qual è la condizione delle zone terremotate delle Marche: lì non si è mosso un mattone. Al di là degli annunci (un miliardo di qua e un miliardo di là) non c'è ancora una lira a disposizione, non vengono pagati i fornitori, non viene pagato nessuno. Qui bisogna agire. La gente è stanca e voi non potete portare portare le persone all'esasperazione. Signora Presidente, intervengo sulla questione che è stata posta da più parti, in particolare da Sinistra Italiana e dal Movimento Democratici e Progressisti, circa la correttezza costituzionale del modo in cui il Parlamento sta procedendo alla ridefinizione della disciplina del lavoro occasionale. Mi sia consentito di osservare preliminarmente che un grave profilo di incostituzionalità sarebbe ravvisabile non tanto nel fatto che il lavoro occasionale venga ridisciplinato, quanto semmai nell'ipotesi in cui esso rimanesse privo di una disciplina adeguata. La Costituzione, all'articolo 35, impone alla Repubblica di tutelare «il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni»: non sarebbe dunque consentito che l'ordinamento, omettendo qualsiasi disciplina della materia, rendesse di fatto impossibile l'incontro fra domanda e offerta in questo specifico segmento, se non nella forma del lavoro occasionale Perché - non dimentichiamolo - il lavoro occasionale autonomo è tuttora riconosciuto dalla disciplina previdenziale e tributaria e non è soggetto ad alcun limite, salvo quello dei 5.000 euro di reddito annui. Vorrei, dunque, chiedere ai colleghi Lo Moro, Barozzino, Cioffi e a tutti gli altri che in questa discussione hanno tuonato contro la nuova disciplina della materia introdotta con l'emendamento aggiuntivo a questo decreto-legge: ma voi volete, dunque, che vengano assunti solo come collaboratori occasionali autonomi (se non addirittura in nero), senza alcuna protezione previdenziale o di altro genere? Ad esempio, i ragazzi ingaggiati la domenica per fare gli assistenti allo stadio prima, durante e dopo la partita, le *hostess* per un congresso, i camerieri per un banchetto, i commessi assunti in un negozio per le due settimane pre-natalizie nelle quali le vendite si triplicano. Sono tutti rapporti che durano poche ore o pochi giorni e, dunque, non sopportano il costo degli adempimenti previsti per il lavoro stabile regolare: raccolta dei documenti personali della persona interessata, apertura di una posizione INPS e INAIL, iscrizione nel libro paga e matricola, redazione e consegna di una lettera con tutti i crismi, comunicazione di costituzione del rapporto alla Direzione territoriale del lavoro competente; per poi ripetere tutte queste operazioni all'inverso all'atto della cessazione del rapporto, poche ore o due giorni dopo. Per il lavoro occasionale subordinato, anche quando ad avvalersene sono le imprese, questi costi di transazione diventano un ostacolo insormontabile, un vero e proprio diaframma che impedisce l'incontro regolare tra domanda e offerta nel campo del lavoro subordinato. Dunque, un sostanziale divieto. Dobbiamo lasciarci alle spalle l'idea sciagurata secondo cui la semplificazione degli adempimenti toglierebbe di per sé dignità al lavoro, così come l'idea che sia socialmente più pericoloso l'abuso commesso in un caso su cento rispetto a una norma che, per evitare quell'abuso, riduca di fatto sensibilmente la possibilità di incontro fra domanda e offerta negli altri novantanove casi. Ma torniamo alla questione di metodo. Tutti sappiamo che, quando il *referendum* viene indetto su materie complesse come questa che non si prestano a essere risolte con un taglio netto, la funzione positiva dell'indizione del *referendum* può attuarsi...

la vecchia disciplina nel senso voluto dai promotori del *referendum*. Questo già avvenne nel 1982, per rimanere sulla materia del lavoro, nel caso del *referendum* sul trattamento di fine rapporto, e nel 1990, con la legge sui licenziamenti nelle imprese di In entrambi i casi, la modifica apportata e ritenuta idonea a evitare il *referendum* fu molto meno incisiva di quella che è oggi al nostro esame. Questo è il quesito che ci dobbiamo porre sulla legittimità sostanziale della modifica di cui stiamo discutendo. Prima di questa modifica i buoni lavoro erano utilizzabili da parte di qualsiasi soggetto e, di fatto, i cinque sesti dei buoni venivano usati da imprese di dimensioni medio-grandi; la soluzione prospettata esclude quasi tutte le imprese, cioè tutte quelle con più di cinque dipendenti. Prima era di fatto possibile l'abuso dei buoni per pagare gli straordinari ai dipendenti regolari o allungarne l'orario effettivo; ora si prospetta un meccanismo che lo rende del tutto impossibile. Il tetto massimo viene abbassato da 7.000 a 5.000 euro l'anno e a 2.500 euro per singolo lavoratore e, al fine di garantirne la piena tracciabilità, ogni pagamento ora deve avvenire per via telematica, a costo di dotare il lavoratore ingaggiato di una carta prepagata.

Se una critica sul piano della costituzionalità può essere mossa a questo nuovo intervento è che esso interviene in modo drasticamente incisivo, al punto da sottrarre alla totalità delle imprese di dimensioni più che minime la possibilità di far fronte alle esigenze di lavoro occasionale

Senatore Ceroni, tutti i colleghi che l'hanno preceduta hanno avuto un paio di minuti in più di quelli contingentati. Lei ha reagito non al mio intervento, ma alla lucetta che lampeggiava; si è inalberato e a quel punto poi ha concluso nei limiti previsti. Se lei fosse andato avanti pianamente, io l'avrei sollecitata e le avrei concesso di parlare due minuti in più. Quindi la inviterei, la prossima volta, a non inalberarsi quando vede la lucetta e ad affidarsi e ad affidarsi alla Presidenza, che cerca di contemperare il contingentamento con le esigenze di ogni oratore di concludere un concetto. Questo glielo consiglio per la prossima volta.

fai una legge di stabilità e la usi come specchietto per le allodole per portare a casa un risultato referendario, prima o poi - come recita il proverbio E oggi paghiamo i conti. Anche laddove sembra che piovano soldi in realtà scopriamo che si tratta, né più né meno, della famosa *gag*: se mi presti dieci euro, ti rendo i dieci euro che mi hai prestato ieri. Vi spiego il perché: perché: ad esempio, all'articolo 22, comma 7-*ter*, è previsto lo stanziamento di cinque milioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale: bellissimo, applausi. La copertura prevede però una riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'assunzione a tempo indeterminato dei famosi 500 funzionari per il Ministero dei beni e delle attività culturali. Anche qui dobbiamo fare a capirci: i funzionari non li assumiamo più a tempo indeterminato o forse sovrastimavamo quei soldi? Bah. Sempre articolo 22, commi 7*-quater* e 7-*quinquies*: al comma 7-*quater* viene istituito uno specifico fondo per il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali. Che bello! Valorizziamo

il coordinamento di tutte le attività per la ricostruzione dei beni artistici lesionati durante i tragici sismi avvenuti lo scorso anno e anche all'inizio di quest'anno, ma la copertura per istituire questo organo dirigenziale viene individuata riducendo l'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore archivi archivi e biblioteche. Anche qui dobbiamo deciderci: la lettura la vogliamo promuovere e valorizzare o no? Sono due esempi e ne potrei portare altri, ma il tempo è tiranno. Mi addentro ora nelle pieghe della manovrina per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali. Per quanto riguarda l'AFAM, l'Alta formazione artistica e musicale, vi risparmio tutta la vicenda che ha dell'incredibile, per non dire del tragico, perché oggi ci ritroviamo ad avere una norma che avrebbe l'ambizione di portare finalmente alla statizzazione degli ex licei musicali e quindi sanare le problematiche legate a questi istituti; peccato però che questa norma, a differenza di un disegno di legge che ancora marcisce in Commissione al Senato, forse dal 2014, è è una norma generica, non prevedendo infatti i termini per l'emanazione dei decreti ministeriali, cioè quelli che dovranno poi descrivere come si dovrà fare questa statizzazione, secondo quali criteri e con quale procedimento. non individua nemmeno le modalità di questa gradualità e quali saranno quindi i criteri per cui si statizzeranno prima certi istituti piuttosto che altri (magari in base alla simpatia del sindaco, non si sa). norma prevede addirittura la razionalizzazione, e noi ormai, in quattro anni di legislatura, abbiamo capito che quando si parla di razionalizzazione si parla di tagli. Questo non era previsto nel disegno di legge dedicato a questo procedimento. In più da dove sono prelevati i fondi? Dai soldi destinati alla ricerca di base, dalle accademie non statali e anche dai fondi che erano stati destinati alla legge sulla buona scuola, con buona pace del segretario PD Renzi e della ex ministra Giannini.

Vi è poi l'ennesima proroga dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari in quelle Regioni in cui è stata risolta la convenzione con la Consip. allo scadere di ogni rinnovo e di ogni proroga, abbiamo detto come l'esternalizzazione non produca alcun risparmio e come, anzi, produca un aumento della precarizzazione sia nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sia nei lavoratori socialmente utili, e come legate alla Consip ci siano alla Consip ci siano inchieste che sono finite anche nel filone della scuola, come quella del 2012 che riguarda un presunto cartello per dividersi un appalto di 1,6 miliardi. Per i beni e le attività culturali dico solo due cose. Per il Teatro Eliseo abbiamo introdotto il metodo Marchionne della contrattazione privata: se conosci il ministro giusto puoi contrattare sui soldi. Evviva! M5S)*. Senza nulla togliere al Teatro Eliseo, abbiamo introdotto il metodo della contrattazione e intanto i teatri in Italia arrancano. In secondo luogo, me lo lasci dire

lede i principi costituzionali della separazione dei poteri; lede il diritto di difesa per i procedimenti in corso. Credo che si sarebbe potuto fare molto di più e molto meglio se, se, *illo tempore*, come sempre, la legge di stabilità non fosse stata utilizzata per delle marchette. Pregherei, nei limiti del possibile, di usare un linguaggio adeguato all'Aula del Senato. Non mi risulta che quella che avete usato in vari interventi sia

Grazie molte manifestazioni da parte dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale perché, con un emendamento parlamentare alla Camera, nell'articolo 27 che citavo all'inizio è stata prevista l'abrogazione del regio decreto dell'8 gennaio 1931, gennaio 1931, n. 148, che - per semplificare a tutti coloro che non lo dovessero conoscere - è l'architrave che ha retto i rapporti all'interno del sistema del trasporto pubblico locale. È una norma cui naturalmente i lavoratori sono molto legati, ma è anche una norma che ha ormai più di ottant'anni. Questa scelta, che personalmente - ma credo di non essere il solo - ritengo sbagliata, è stata inserita, come dicevo, attraverso un emendamento. Teniamo conto che siamo in una fase molto rilevante per il trasporto pubblico locale, perché in molte Regioni stanno partendo le gare per l'affidamento del servizio. regio decreto n. 148 sono contenute alcune norme di salvaguardia, in particolare la clausola sociale, che che tutela naturalmente i lavoratori nel caso in cui vi fosse un cambio di appalto e voi capite che, essendo questo l'anno in cui comincia davvero la liberalizzazione del

di essere attualizzato: occorreva verificare quali norme erano ancora attuali e quali avrebbero richiesto, invece, una revisione. Dopo l'approvazione alla Camera, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministro Delrio, si è avviato immediatamente un tavolo con alcuni sindacati più importanti e rappresentativi (CGIL, CISL, UIL, FAISA e UGL), che ha portato, nella giornata del 12 giugno, alla sottoscrizione di un verbale di accordo per cercare di indirizzare un percorso a fronte di questa abrogazione. abrogazione. Visto e considerato che la norma prevede un anno di tempo per i sindacati e le associazioni datoriali per recuperare, all'interno del contratto collettivo nazionale,

di tutela, ad esempio sul tema della clausola sociale, quella più rilevante, in caso di cambio appalto. Faccio allora una richiesta al Governo, qui rappresentato dal vice ministro Morando: credo che il verbale di accordo sottoscritto dal ministro Delrio con i sindacati sia un importante strumento di lavoro,

venga accompagnato da una cornice legislativa. Lo dico perché su questo terreno ci sono state molte polemiche e alcuni colleghi in quest'Aula hanno richiamato questa soppressione come un tentativo di sottrarre diritti ai lavoratori. Faccio presente che gli stessi sindacati - molti di loro

mesi di tempo solo alle organizzazioni sindacali, ma che si coinvolgano pienamente l'Esecutivo e il Parlamento nell'azione di costruzione di una cornice, in modo che non ci siano dubbi sulla volontà, da parte del Parlamento, del Parlamento, di accompagnare un processo serio, di revisione di una norma che ha garantito, in questi oltre ottanta anni, il funzionamento e la tutela dei lavoratori del sistema del trasporto pubblico locale. PRESIDENTE. Signora Presidente, oggi ci troviamo a discutere della cosiddetta manovrina, ovvero dell'adeguamento della legge di bilancio alle indicazioni della Commissione europea. al solito le promesse da marinaio, ovvero le chiacchiere del DEF e i numeri fantasiosi della legge bilancio, ci rendono la solita figura da Pinocchio. Sono serena, per carità - di nome e di fatto - e vorrei anche credere con fiducia a quanto detto dal ministro Padoan, che ci prospetta una crescita po' miope - non riesco ad andare oltre la situazione critica in cui versa l'economia reale, quella dei tanti imprenditori e liberi professionisti, che sono vessati da mille emendamenti

Mi riferisco in particolare allo *split payment*, nato con l'intento di ridurre l'evasione fiscale, per aumentare il gettito a favore dello Stato, che rappresenta però, di fatto, non una pioggia sul bagnato, ma una grandine che distrugge ciò che di sano nella nostra economia reale è rimasto. La pubblica amministrazione è il peggior cliente che imprese e professionisti possano avere. Signori miei, lo *split payment* uccide le imprese. Imprenditori e professionisti già devono pagare in anticipo il 20 per cento dell' IRPEF, con il meccanismo della ritenuta d'acconto e hanno l'obbligo della fatturazione elettronica, con la nuova trasmissione trimestrale dell'IVA, con tanto di vessazione dello spesometro, introdotta proprio per avere uno strumento antievasione, perché in questo modo si tracciano tutti i compensi ricevuti. In tal modo siamo diventati tutti Bancomat di uno Stato inadempiente ed inefficiente. Lo *split payment* altro non è che un finanziamento forzoso allo Stato da parte di privati, imprese e professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione. Ma non contento, lo Stato, sempre con il suo stile burocratese e assurdo, prova a metterci una pezza che è peggio del buco. Noi abbiamo sostituito l'efficienza e la preparazione dell'ENA francese, che sforna politici illuminati che vanno verso la deregolamentazione, la semplificazione e l'apertura, con una laurea che sembra data dall'"ufficio complicazioni cose semplici". Ulteriore burocrazia che consiste nel dover chiedere allo Stato quanto mi è dovuto, con annessi costi da parte di privati e della stessa Agenzia delle entrate: l'amministrazione è così complicata e contorta che complica la vita ai privati cittadini, ma se la complica essa stessa; il tutto in tempi che vanno dai sei mesi ai due anni. Inoltre, lo *split payment* mette in conflitto imprenditori, professionisti e imprese che vantino un credito di IVA di tipo ordinario nei confronti dello Stato e quelli che sono obbligati dalla legge ad avere un credito IVA. Si genera una competizione tra privati per vedere garantito un proprio legittimo diritto. La logica vorrebbe che, in tutti i casi in cui sostituisce un automatismo d'imposta con una nuova procedura, questa sia più efficiente e renda l'attività di impresa più facile. Invece cosa è successo? Il Governo, lungi dal risolvere un problema esistente, estende questo meccanismo a tutte le imprese e i professionisti, sottoponendoli a un'inutile e dannosa barbarie. Quello che avreste dovuto fare, urgentemente, era una cosa sola: estendere il pagamento dell'IVA per cassa a a tutte le categorie, risolvendo così tutti i problemi collegati e aumentando davvero il PIL. Perché quando si rende certezza della legge, quando le attese sono chiare e soddisfatte, c'è anche una propensione automatica ad investire e fare impresa. Ma se, da un lato, al fine di reperire risorse, si trovano soluzioni aberranti e dannose per le imprese, dall'altro ben sappiamo come impiegarle; è sconcertante come in questo decreto-legge, da un lato, si sposti il peso della manovra sulle imprese già massacrate dalla crisi e senza liquidità e, dall'altro, si foraggi il lusso e il superfluo. Anche in questa manovra il Governo ha reinserito un premuroso pensiero alla Ryder Cup 2022, come già tentato nel milleproroghe e nel disegno guarda caso, tutti provvedimenti che passano con la fiducia e non attraverso il confronto. L'articolo 63 prevede la concessione di 97 milioni di euro a favore della Ryder Cup Europe, Cup Europe, che si aggiungono alla quota già stanziata dalla legge di bilancio 2017. I contribuenti pagano e ripagano: prima la parte pubblica, ora la garanzia per gli investimenti privati. Io capisco che le banche abbiano bisogno di garanzie; capisco che devono essere molto oculate, ma devo essere io cittadino ad assicurarle? Io che, quando vado in banca e chiedo un prestito, trovo sempre la porta chiusa? Io devo garantire la banca? Noi vincoliamo in questo momento 97 milioni che lo Stato avrebbe potuto rivolgere verso esigenze davvero urgenti e davvero indifferibili. Vi ricordo il terremoto, che sta ancora tutto là. A proposito del terremoto, l'unico aspetto positivo di questo decreto-legge è l'istituzione di zone franche urbane, che io sinceramente ho sollecitato più volte. Addirittura sono depositati diversi disegni di legge che bastava copiare, ma neanche quello è stato fatto, perché anche in questo provvedimento si è riusciti a fare una norma totalmente avulsa dalla realtà; una norma che non tiene conto di come va l'economia e del Paese, e non ha considerato nessun suggerimento. Mi chiedo come si possa pensare di istituire una zona franca urbana, che in quest'Aula è stata sollecitata più volte anche dalla sottoscritta già dallo scorso dicembre, che preveda dei benefici fiscali - ascoltate bene

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. Vi ricordo che il terremoto è avvenuto ad agosto ma è ovvio che i danni del terremoto non possono essere limitati al 2016 e vanno avanti. Tutto rispetto al corrispettivo periodo del 2015: sarebbe stato utile, giusto e congruo un confronto ma non con un periodo di tempo così limitato e non in questi termini. Questa formulazione equivale, di fatto, a non concedere il beneficio a nessuno e ad assicurare l'evasione fiscale per qualcuno che magari ci prova. Per non parlare del fatto che le agevolazioni sono concesse per soli due anni, due anni, ma un investimento, se il sollievo è di soli due anni, non trova ristoro quando vai a confrontarti con una realtà già provata e difficoltosa in partenza.

perché possono campare solo di politica e non sanno cosa vuol dire fare impresa, non sanno cosa significa lavorare, non sanno cos'è la vita reale. in questo provvedimento mi preme sottolineare una questione ricorrente che si Grazie

lavori pubblici, abbiamo avuto l'audizione dei commissari di Alitalia e devo dire che sta venendo fuori quello che da diverso tempo noi sottolineavamo al Governo - in questo caso al ministro Delrio e non solo

All'interno di questa manovra, mancano le azioni che dovrebbero, in questo momento di difficoltà rafforzare e rimpinguare, non solo sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto gestionale di presenza della politica all'interno di questa importante partita delle infrastrutture e dei trasporti; ciò è del tutto evidente.

la questione del passaggio di ANAS all'interno del gruppo FS, la questione della modifica del codice degli appalti, l'annosa questione che sottolineava prima un collega del della messa in sicurezza di un tratto autostradale strategico nel nostro Paese che è l'A24 e l'A25. Come si dice dalle mie parti, si evince chiaramente che manca il manico, da questo punto di vista.

doveva arrivare un altro fenomeno come Gubitosi (che alla Rai è stato bravissimo, dal mio punto di vista) per dire che, in due giorni, cambiando lo Statuto, potevamo essere competitivi con Ryanair e *company* e sfidarle sullo stesso terreno? Collega Morando,

Grazie

alla pari con i nostri *partner* europei. Ben diverso è invece il sistema di trasporto ferroviario locale, che dovrebbe essere implementato per numerosissimi

sulla base di dati oggettivi ed inconfutabili. In pochi giorni, il Governo italiano ha ricevuto due ambiti riconoscimenti da parte dell'Istat e del Fondo monetario internazionale, entrambi convinti che la crescita, almeno per il 2017, sarà leggermente superiore a quella prevista dai documenti del Ministero dell'economia. Ed è bastato questo per brindare, dopo aver tirato un sospiro di sollievo. Purtroppo in Italia abbiamo la cattiva abitudine di soffermarci solo sui titoli e di non leggere il contenuto degli articoli, un po' come in quel vecchio proverbio cinese cui lo stolto si ferma a guardare il dito che indica la luna e non guarda la luna. Applicare questo metodo ai ponderosi documenti programmatici rischia di giocarci un brutto tiro di farci scambiare lucciole per lanterne: le dichiarazioni conclusive dello *staff* che ha terminato la sua missione in Italia ai sensi, vice ministro Morando, dell'*Article* *IV* del Regolamento del FMI, sono molto più caute di quanto riportato dalla stampa italiana (che spesso mette dei titoli per vendere i giornali e il contenuto dell'articolo è diametralmente opposto

Nel dettaglio: «incoraggiate dai dati del primo trimestre, le proiezioni per quest'anno sono dell'1,3 per cento circa. Poiché i venti a favore - condizioni commerciali, politiche fiscali e monetarie - diverranno meno

La crescita potrebbe sorprendere in positivo nel breve periodo, sulla scia di una più forte ripresa a livello europeo. Tuttavia, i rischi di ribasso sono significativi, correlati tra l'altro a fragilità finanziarie, incertezze politiche, eventuali battute d'arresto al processo di riforma» - ovviamente in questi ultimi mesi non si di riforme, il nostro Gruppo era nato per sostenere quelle riforme, ma non siamo in grado di farlo perché non ce ne sono più - «ed a revisioni della valutazione dei rischi di credito nell'ambito della normalizzazione della politica monetaria». delle conclusioni dello *staff* del Fondo monetario internazionale. Questo è quindi il quadro completo. Va bene che in Italia siamo abituati all'ottimismo della volontà. Esso andrebbe, tuttavia, compensato dal pessimismo della ragione, o almeno dal suo necessario realismo, di cui purtroppo non si vede traccia nelle dichiarazioni dei nostri Ministri responsabili o irresponsabili. Del resto, forse per un eccessivo senso del pudore, le previsioni di più lungo periodo del Fondo sono state un po' come il responso della Sibilla.

sostengono infatti che il reddito *pro capite* dovrebbe tornare a livelli pre-crisi solo tra qualche anno e che l'Italia divergerebbe ulteriormente dai pari dell'eurozona: è un disastro, sentenza poco rassicurante. Il Governatore della Banca d'Italia nelle sue ultime considerazioni finali di pochi giorni fa

Quindi abbiamo ancora dieci anni per tornare al PIL del 2007 e nel frattempo che fine faranno i nostri giovani già costretti a sobbarcarsi dell'onere maggiore della crisi e quei poveri che continuano aumentare continuamente, come ci dice l'ISTAT, e le tante famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese? Potrei continuare all'infinito, ma questa è demagogia, falso populismo. Non illudetevi quindi, colleghi, signori rappresentanti del Governo, e soprattutto non illudete gli italiani. La coda è sempre la parte più difficile da scorticare e certe manifestazioni rassicuranti non sono altro che uno schiaffo alla miseria. Tutti i vostri ragionamenti sono fondati sugli ultimi dati Istat, che ha rivisto al rialzo le stime del primo trimestre da un iniziale 0,2 allo 0,4 Già su questo balzo improvviso si potrebbe eccepire: una correzione del 100 per cento non è un fatto usuale, non è normale, c'è qualcosa che non va: non si può sbagliare del 100

quella maggior crescita deriva solo dall'accumulo delle scorte, niente di più. I nostri industriali, i nostri imprenditori hanno prodotto e messo nei magazzini

(elettroencefalogramma piatto): fermi i consumi, immobili gli investimenti, la domanda estera che tira sempre meno, gli imprenditori dall'estero che non vengono in Italia perché non si fidano della nostra burocrazia e della nostra malagiustizia.

con fiducia viene ad investire in Italia. Sono sempre meno. Nella fisiologia del ciclo economico la variabile "scorte" è sempre il dato più volatile. Il relativo accumulo può derivare da due elementi contrapposti: una maggior fiducia delle imprese che producono per il magazzino nella speranza (che è l'ultima a morire) che i consumi possano riprendere, oppure sono la risultante di una domanda cresciuta meno del previsto. Per concludere, signora Presidente, su questo dato così labile, come abbiamo visto nel testo licenziato dal Fondo monetario internazionale, si costruiscono scenari iperbolici. Dobbiamo, invece, rimanere con i piedi per terra. Grazie a questo esercizio di umiltà è possibile vedere come realmente stanno le cosa e approntare, pure nella ristrettezza dei tempi che ci consegna questa legislatura, le possibili risposte. Un testimone da consegnare al futuro Governo nel prossimo anno, all'indomani delle elezioni. Ci vuole più coraggio, ma anche un po' di capacità. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la manovra prova quanto il Governo abbia fallito con la legge di stabilità del 2017, quanto la situazione si sia fossilizzata in perdita e quanto l'Italia non sia altro che una mera colonia alle dipendenze di ordini che arrivano dall'alto. Non solo siamo alla mercé degli ordini europei, ma non siamo neanche capaci di rispondere in maniera adeguata. Stiamo sempre a sottolineare che la situazione cambierà negli anni successivi: sempre l'anno dopo, mai quello attuale. Si vorrebbe tamponare il buco esistente basandosi soprattutto sulla lotta all'evasione fiscale; una lotta che in tal modo viene presa in considerazione solo quando c'è da rinsaldare qualche conto, solo a botte di condoni. Da Renzi a Gentiloni Silveri il copione non è cambiato, un contrasto che resta sulla carta, del tutto asistematico. Basti pensare al fatto che benché tra Governo Renzi e Governo Gentiloni Silveri il tema evasione sia stato toccato per ben otto volte, la somma che il fisco, a partire dal 2015, è riuscita a farsi restituire è diminuita, così com'è testimoniato nella relazione della Corte dei conti. Allo stesso modo si parla di riduzione del numero di apparecchi per il gioco, ma non c'è nessuna disposizione specifica che punti, nel lungo periodo, a destabilizzare la *lobby* dell'azzardo e a prevenire a monte il gravissimo problema sociale della ludopatia, che ormai affligge la nostra società; vengono sempre e solo ipotizzate irregolarità da sanare. L'Italia continua a essere stretta nella morsa del «ce lo chiede l'Europa» e delle solite correzioni dei conti pubblici per non appesantire ulteriormente l'indebitamento. È la solita truffa del debito pubblico, quando l'unico vero inconveniente è dato dal fatto che lo Stato è diventato succube della finanza privata e la BCE può garantire privilegi sugli interessi soltanto alle banche private e non agli Stati che, per forza di cose, possono solo «tirare a campare», tagliando servizi essenziali e cercando di rattoppare, nel breve periodo, quel tanto che basti per non cadere nel baratro più profondo. Questi ultimi Governi non hanno fatto altro che incentivare la subordinazione della politica a una oligarchia finanziaria mettendo sempre più alla sbarra la partecipazione diretta dei cittadini, che rimangono inermi spettatori spettatori che devono sperare, anno dopo anno, di sfangarla, vuoi a causa delle clausole di salvaguardia (il cui impatto è comunque soltanto leggermente ridotto), vuoi per l'incremento delle accise e simili. È inutile dire che ci si è concentrati sulle partite IVA perché, pur non aumentando formalmente la pressione fiscale, la situazione non cambia e in Italia è impossibile produrre. Fare impresa per i giovani, per coloro che non dispongono di ingenti capitali (quelli incamerano semplicemente fondi pubblici e poi delocalizzano a spese dei lavoratori) significa sempre e ancora dare allo Stato, a conti fatti, oltre il 50 per cento di ciò che si dichiara, senza alcuna tutela che possa riparare dalla crisi dilagante. Vediamo solo misure estemporanee, quel tanto che basta per non compromettere troppo l'esito delle future elezioni, per riuscire a tenere almeno la testa fuori dall'acqua. Intanto, illustrando il 25° rapporto sui cambiamenti economici, i dati Istat ci dicono che oltre 7 milioni di persone vivono in grave deprivazione materiale e per gli *under* 35 è sempre più difficile trovare lavoro. viene compiuta in materia di diseguaglianza sociale, considerando che la spesa per consumi delle famiglie ricche è più che doppia rispetto alle famiglie a basso reddito e che sempre un numero maggiore di italiani rinuncia alle cure mediche per mancanza di soldi. Lo stesso rapporto Istat tra l'altro spiega che "la capacità redistributiva dell'intervento pubblico è in Italia tra le più basse d'Europa". Nessun provvedimento mirato e di largo respiro in materia di politica industriale: si va sempre più verso la desertificazione, una desertificazione che porta via con sé milioni di lavoratori. E nel frattempo si prospetta la ratificazione di accordi, promossi in seno all'Unione europea, che si rendono sempre più portatori

Si tende a fare in modo che i privilegi delle grandi multinazionali abbiano una via privilegiata, addirittura di natura legale, preordinata ai bisogni e alle necessità del popolo. I lavoratori non hanno bisogno di ulteriori vostre prese in giro: si può cambiare anche il nome ma il risultato di contratti che stralciano ogni diritto duramente conquistato in anni di lotte, senza vedersi riconosciute ferie, malattie e infortuni, non fa onore a nessuno: anzi. Servono provvedimenti per far si che si possa prospettare un futuro per questo Paese, che appare sempre più disorientato da una orda neoliberista, senza prospettare in continuazione speranze vane e mettendo da parte le mosse strategiche dettate solo dalle esigenze elettorali. *(Applausi del Presidente, noi vogliamo esprimere il nostro pensiero sul merito di questa manovra che, lo dico senza alcun problema, noi sosterremo, anche con il voto di fiducia. non perché sia un provvedimento che rilancia l'economia del Paese, in quanto ha un limite, che è quello dato dall'oggettività della sua funzione principale: quella di intervenire in corso di esercizio anche ad adempiere ad obblighi di natura internazionali che ci siamo dati e che si esplicitano all'interno dei nostri provvedimenti in materia di finanzia pubblica dentro uno schema, che che è quello che condividiamo e che per fortuna c'è; altrimenti, molti Paesi europei avrebbero pagato prezzi molto più salati di quelli che hanno pagato sul fronte della crisi:

che questa manovra cerca di soddisfare, quindi anche evitando eventuali problemi di natura sanzionatoria. Lamentiamo una cosa, che credo sia stata lamentata da tutti, per primi dai componenti della Commissione bilancio: il fatto che

perfetto, dove Camera e Senato hanno tutti e due il diritto/dovere di intervenire sulla definizione dei provvedimenti. però, alcune esigenze che noi abbiamo ritenuto importanti soprattutto per quanto riguarda le zone colpite da recenti calamità naturali, in quanto cerca di rimediare a una situazione di emergenza. Non è sufficiente. Abbiamo proposto ordini del giorno che integrano questo tipo di intervento e che cercano di rimediare alle condizioni di difficoltà delle Province italiane. Le Province devono continuare ad esercitare le proprie funzioni fondamentali in segmenti importanti, come quelli della viabilità e dell'istruzione. altro punto; lo dico perché parlo anche per esperienza professionale diretta. Per fortuna, anche se il Governo lo sa e avrebbe potuto fare passaggi di dialogo con le forze sociali delle imprese e del lavoro prima di definire il provvedimento, lo stesso interviene a regolare il lavoro occasionale in modo puntuale e io credo anche molto restrittivo, rispondendo a quelle che erano state le esigenze poste dalla grande mobilitazione in materia di abrogazione delle disposizioni sui *voucher*, per contrastare l'abuso di uno strumento e di un istituto come questo e non per cancellarne la funzione, che invece è indispensabile. Noi vogliamo una regolazione severa e un controllo diretto e continuo sull'applicazione dell'istituto, ma il lavoro occasionale è un lavoro che esiste e che va regolato; quindi bisogna prendere atto di questa esigenza. Va regolato e controllato, perché l'abuso sia definitivamente cancellato. Dopodiché questa è anche un'occasione per fare un ragionamento politico di carattere generale, rispetto alla responsabilità che tutti noi abbiamo nei confronti del Paese, e anche un'analisi dell'umore che il Paese esprime. Io credo che non ci sia alternativa di Governo democratico in questo Paese che non sia il centrosinistra; questo è un pensiero che condivido con diversi senatori che stanno con me in questo Senato a vivere un'esperienza di costruzione del centrosinistra partendo dall'iniziativa di Campo Progressista. Campo Progressista è un progetto di unità del centrosinistra che meglio si sostanzia proprio in queste circostanze. Noi sosteniamo il Governo

si vada a votare in sicurezza democratica, possibilmente con un insieme di regole che rispettino i principi costituzionali di rappresentanza e governabilità. E in questo quadro noi riteniamo irrinunciabile il confronto con tutte le forze politiche e sociali del centrosinistra, a iniziare dal Partito Democratico, che è per noi un alleato solido in tante situazioni che abbiamo affrontato e che affrontiamo positivamente nelle difficili prove di governo in Regioni, territori e città. con il Partito Democratico ci siamo presentati e ci presentiamo anche in questi giorni a chiedere il consenso agli elettori. Noi sentiamo la missione per il rafforzamento del centrosinistra, anche assumendoci questa responsabilità di voto come irrinunciabile per assicurare al Paese le necessarie capacità ad affrontare i gravi problemi dell'economia e della società italiane. Siamo consapevoli della necessità di superare i limiti di coesione e di efficienza politica del centrosinistra; pensiamo però che il centrosinistra, con il Partito Democratico, rimanga l'unica risposta politica vera ai bisogni e alle difficoltà di vita delle persone, soprattutto di quelle in maggiore sofferenza e marginalizzate, e l'unica risposta alle esigenze crescenti delle nostre comunità più fragili. Al contempo è una giusta risposta di contrasto alle derive populiste, xenofobe e autoritarie che ci sono in Italia, in Europa e nel mondo. Per questo sentiamo l'esigenza di una nuova, articolata e unitaria proposta politica. È chiaro che di centrosinistra in Italia ne esiste uno solo, non ce ne sono tre o quattro, perché i conti ce lo dicono: è quello della buona combinazione tra il Partito Democratico e le forze di sinistra con cultura di governo e che si rendono disponibili a un percorso comune. Noi abbiamo assunto questo impegno e intendiamo mantenerlo. Certo che aiuterebbe molto capire se questa volontà ci sia anche nel Partito Democratico in ogni circostanza, senza strumentalità. Siamo in questo però, per quanto ci riguarda, assolutamente coerenti anche nell'aver condiviso con Giuliano Pisapia la positiva evoluzione dell'esperienza di governo del centrosinistra in tanti Comuni e Regioni d'Italia, da Cagliari a Milano, dalla Puglia al Lazio. Voteremo la manovra, quindi, non solo per un ragionamento di merito, ma anche per un ragionamento politico. Signora Presidente, oggi porto in questa Assemblea innanzitutto la voce di 83.000 studenti degli istituti scolastici, dei loro genitori e di tutti lavoratori della Provincia di Caserta. Vorrei innanzitutto illustrarvi l'attuale situazione: non so se volontariamente o involontariamente, il Governo ha sottovalutato fino a oggi la grave situazione che il dissesto della Provincia di Caserta sta causando e che a breve porterà a un totale collasso a cui sarà probabilmente impossibile porre rimedio. È vero, sono tante le Province in difficoltà, ma Caserta rappresenta forse la situazione più grave. È più di un anno che con interrogazioni, emendamenti in vari provvedimenti, note e solleciti in Aula stiamo denunciando il lento declino di una Provincia intera. E non si faccia l'errore di interpretare la parola «provincia» solo come ente locale. Dobbiamo pensare soprattutto alla popolazione di quella Provincia che per prima subisce disagi di una cattiva e in questo caso assente gestione ordinaria. Tutto quanto sino ad oggi, già da noi denunciato, purtroppo è rimasto lettera morta. Allora voglio spiegarvi qual è la reale situazione e quale la soluzione che vi stiamo proponendo. Sappiamo già tutti che verrà posta la questione di fiducia, ma ho la necessità e il dovere di parlarvene affinché le nostre denunce rimangano agli atti di questa seduta, perché domani nessuno potrà avere la scusa di dire di aver fatto il possibile, perché così non è stato. La Provincia di Caserta ha dichiarato il dissesto a dicembre 2015. Questo ha comportato l'impossibilità di approvare il bilancio previsionale 2016 e l'impossibilità di qualsiasi azione che comportasse movimenti di cassa: quindi *stop* a manutenzione a scuole e strade, *stop* a stipendi dei dipendenti, *stop* alla gestione dei beni culturali di propria competenza. A Caserta ci sono 93 istituti che fanno capo alla Provincia con circa 83.000 studenti. A fine anno 2016 alcuni istituti sono stati chiusi perché a rischio crolli. A maggio un altro istituto, il Buonarroti, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri per lo stesso motivo. Essendo il 90 per cento di questi istituti non a norma, per ciò che riguarda le certificazioni per la sicurezza, probabilmente non potranno aprire per il nuovo anno scolastico questo sarebbe un danno enorme per gli 83.000 ragazzi che perderanno un anno di studi. Questo perché la Provincia ha dato lo *stop* a tutte le attività di manutenzione e addirittura di erogazione di energia elettrica e riscaldamento, oltre all'aver interdetto gli istituti tecnici all'utilizzo dei laboratori. La stessa situazione vale per le strade: lo *stop* ovviamente ha riguardato anche la manutenzione delle strade provinciali, con tutte le conseguenze immaginabili per rischio di incidenti e incolumità dei cittadini tutti. Anche i beni culturali stanno andando in rovina: ci sono musei, come il Museo campano di Capua, che sta cercando di resistere, ma che rischia la chiusura perché la Provincia non può provvedere alla più minima azione di gestione. un museo su tre piani, grandissimo, straordinario, con reperti unici risalenti al 500 avanti Cristo. I lavoratori della Provincia e delle società da essa dipendenti non percepiscono ormai lo stipendio da tre mesi e la soluzione non si intravede a breve. Quindi ci sono intere famiglie, anche monoreddito, che sono in enorme difficoltà, mentre i lavoratori dell'indotto sono stati già interamente licenziati e mandati a casa. La sede principale della Provincia è ormai chiusa da oltre un mese e mezzo, perché non potendo la Provincia rinnovare il contratto alla società di pulizie, non sono state garantite le condizioni igienico-sanitarie e anche gli uffici, che hanno occupato in via temporanea, domani chiuderanno per lo stesso motivo. Sulla questione scuole si potrebbe rispondere che sono stati stanziati fondi per l'edilizia scolastica, ma se la Provincia non esce dal dissesto non li si potrà utilizzare e i tempi sono strettissimi, visto che a settembre dovrebbe in teoria iniziare il nuovo anno scolastico. Per la questione dei lavoratori, si potrebbe rispondere che sono stati stanziati altri 10 milioni di euro, esclusivamente per le Province in dissesto a dicembre 2015,

Ebbene, per uscire da questa situazione sarebbe stato necessario approvare un emendamento, che abbiamo proposto già in occasione di altri provvedimenti e che abbiamo ripresentato per il decreto-legge in esame, con il quale si intende esonerare dal pagamento del contributo annuale le Province che hanno dichiarato il dissesto finanziario al 31 dicembre 2015. Questo emendamento, considerato che verrà posta la questione di fiducia, è stato trasformato in un ordine del giorno, impegnando il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di esonerare dal concorso al contenimento della spesa pubblica altresì le Province che risultino in stato di dissesto finanziario alla data del 31 dicembre 2015.

Solitamente non mi ritengo molto soddisfatta dell'approvazione degli ordini del giorno, perché raramente si dà seguito all'impegno preso. Devo dire però che le parole del vice ministro Morando mi fanno ben sperare che quanto da me detto in Commissione sia stato ben compreso e che, seppur nel decreto-legge in esame non è possibile inserire nulla, molto probabilmente in seguito il Governo sarà costretto a prendere provvedimenti per la provincia di Caserta, che vanno oltre quanto previsto e inserito nel decreto-legge in esame alla Camera dei deputati. Infatti lei, Vice Ministro, ha dichiarato che, nonostante le misure intraprese alla Camera dei deputati per le Province in dissesto al 31 dicembre 2015 e i fondi stanziati per l'edilizia scolastica, effettivamente, considerata l'eccezionalità della situazione, essi potrebbero non essere utilizzati dalla Provincia di Caserta in quanto, essendo in dissesto, non può effettuare alcuna operazione finanziaria e di cassa. Pertanto ha ammesso che il Governo potrebbe valutare in seguito un'azione, in modo da risolvere questo tipo di intoppo anche, se necessario, attraverso l'esonero del contributo annuale. È questo il motivo per cui avete accolto questi ordini del giorno come impegni e non come raccomandazioni. Avviandomi alla conclusione, detto questo non mi rimane altro che sperare che provvediate prima che sia troppo tardi e - non lo vorrei dire, ma lo devo fare - spero che provvediate prima che si verifichi una tragedia nelle scuole o un atto di disperazione di cittadini privi ormai da mesi dello stipendio. Chi vi sta parlando oggi non è semplicemente una collega di un Gruppo politico avversario: in questo momento chi vi sta parlando è innanzitutto una cittadina casertana che vi riporta il grido di aiuto di una intera Provincia. Vi chiedo di dare ascolto a questo grido.

più significativi, in termini macrofinanziari, della manovra al nostro esame, per svolgere quindi una riflessione di carattere istituzionale, che mi sta molto a cuore.

di euro. Già dal 2018 questa entrata - dice il Governo - comincia ad essere compensata da un minore pagamento di IVA da parte delle imprese o dei lavori autonomi assoggettati allo *split payment*. aggiunge un'enorme nuova entrata, quantificabile anche questa in circa 1,9-2 miliardi, dovuta alle compensazioni indebite che vengono abbassate

riducono di un importo considerevole le clausole di salvaguardia che, com'è noto, farebbero scattare l'aumento dell'IVA. Qual a mio avviso, il grave *vulnus* alle finanze pubbliche che questo sistema certamente certamente produrrà? Noi abbiamo due maggiori entrate importanti di cui una relazione tecnica forse troppo complessa non dà

Sostanzialmente, com'è noto, lo *split payment* prevede che lo Stato, gli enti pubblici, gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali versino immediatamente all'Agenzia delle entrate le imposte che invece avrebbero dovuto pagare alle imprese e da queste poi versate e, al di là del carattere di anticipazione, conferisce loro, a partire dal 2018

per almeno il 2018 e il 2019, che poi si riduce di 500 miliardi dal 2020. Ma vediamo gli anni più vicini. Si sostiene da parte del Governo che,

che non trovi una esauriente dimostrazione da parte del Governo; ritengo inoltre che questa cifra sia esageratamente valutata perché, per un verso,

il possibile minore sviluppo che una simile manovra produce. Spesse volte ci lamentiamo dell'Italia che cresce un po' meno degli altri e penso che queste manovre contribuiscano. Analogamente, a mio avviso è esageratamente valutato il risultato prodotto dalla riduzione della soglia della certificazione per le indebite compensazioni. Parliamo anche in questo caso di cifre assolutamente importanti, nell'ordine di circa 2 miliardi l'anno a partire dal 2018. Non c'è, a mio avviso, un'adeguata dimostrazione, mentre gli effetti sono calcolati precisamente perché essi vengono impiegati per il 2017 per raggiungere un miglioramento dei parametri che ci viene richiesto dall'Unione europea, ma dal 2018 in poi vengono impiegati in maniera puntuale per una grandezza ben nota e ben cifrata che è quella dell'IVA che deve essere aumentata

Se posso aggiungere con una piccola dose di ironia, qualcuno ha detto che sarebbe stata prevista la *web tax* per coprire i minori introiti della Tobin *tax*. Meglio di no, a mio avviso, si sarebbero aggiunti due minori introiti. Ecco, questo è il timore che nutro verso una manovra alla cittadinanza, agli italiani, alle imprese italiane, ai lavoratori autonomi italiani per rientrare nei parametri, cioè per una forma, seppure non eccessiva, di risanamento della finanza pubblica. Essa potrebbe

Con tutto il rispetto che uso dare alla Presidenza del Senato che ha un altissimo rilievo istituzionale, mi permetterò di sottoporle, signora Presidente, una critica molto decisa. Il mio cruccio è che queste domande, e le possibili risposte da parte del Governo, sarebbero state possibili in una una discussione ampia, serrata ma seria, come è sempre costume del Senato in queste discussioni, quale che sia il Governo, quale che sia l'opposizione. Una interlocuzione di questo tipo, su cifre di questo tipo, trova normalmente nel Senato della Repubblica, sia in sede di Commissione che in sede di Assemblea, il suo luogo naturale per esprimersi: ci sono

ha l'obbligo di dire che il Senato della Repubblica deve valutare le manovre finanziarie. Deve avere l'intera prerogativa di emendabilità, di discussione e di miglioramento. Questo, signora Presidente, comincia a diventare un *vulnus* francamente non sopportabile.

la manovra fu adottata a cavallo di una crisi di Governo e, seppur non ritengo sufficiente una crisi di Governo per impedire un dibattito completo - ribadisco le facoltà e le prerogative specie su un provvedimento importante come quello, però non dimentico di essere un parlamentare e, quindi, sono disponibile a comprendere alcune priorità. Capisco che una crisi di Governo è un evento traumatico

alcun elemento che potesse impedire a questo ramo del Parlamento una discussione serena, ampia e approfondita. Signora Presidente, la prego di tener conto di questa mia osservazione perché non si abbia più a vedere una situazione come quella che il Senato sta più volte - troppe volte - ormai insostenibilmente affrontando, ossia non prendere parola in senso concreto - ribadisco, nella pienezza dei suoi poteri - sui provvedimenti di natura finanziaria.

il relatore ha fatto un'esauriente illustrazione dell'intero provvedimento e molti degli interventi che mi hanno preceduto hanno affrontato tantissimi temi. Voglio soffermarmi ad approfondire

di misure molto attese, che in parte hanno recepito le richieste dell'ANCI, dell'UPI e delle Regioni e che sicuramente, per quanto riguarda Comuni e Regioni, hanno completato il quadro già delineato dalla legge di bilancio

si prevede un incremento di 11 milioni di euro per il 2018. Si cerca di contenere gli effetti della perequazione rispetto alle risorse storiche di riferimento, proprio per evitare ai Comuni un impatto troppo brusco nel ridimensionamento dei trasferimenti. Sono stati inoltre concessi dei tempi più ampi per rispettare le regole della nuova contabilità, proprio perché i Comuni si stanno dotando di tutti gli strumenti per affrontare le regole del nuovo regolamento di contabilità, ma alcuni sono ancora in difficoltà. Pertanto, vengono dilazionati i tempi per lo scioglimento dell'ente in caso di mancata approvazione del rendiconto e viene spostata al 31 luglio 2017 la scadenza per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale

un incremento di un milione di euro, per il 2017 e il 2018, del contributo a favore dei Comuni che danno luogo alle fusioni. Anche da questo punto di vista, c'è il tentativo di accompagnare un processo che ormai dura da tempo, ma che

degli aspetti che mettono in maggiore difficoltà gli enti locali, proprio perché riguardano i ragazzi delle proprie comunità e la messa in sicurezza del tempo che questi trascorrono all'interno di queste strutture. Vi sono disposizioni concernenti l'impiego dell'avanzo destinato sempre agli investimenti degli enti locali ed anche per l'estinzione anticipata dei prestiti. che vanno a completare misure già presenti in provvedimenti precedenti e che danno il senso dell'attenzione nei confronti degli enti locali. Anche nei confronti delle Regioni, i provvedimenti individuati sono parecchi e concernono sia il rinvio del ricorso ai fabbisogni *standard* e capacità fiscali delle Regioni, ma anche l'entrata in vigore dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni, il TPL, gli investimenti, prevedendo Tutto ciò crea un quadro favorevole nei confronti di questi livelli assistenziali. Molti articoli riguardano anche le Province e le Città metropolitane, perché sono proprio questi gli enti con maggiori difficoltà. Viene definita la ripartizione del taglio incrementale di 900 milioni in 650 milioni a carico delle Province e 250 milioni a carico delle Città metropolitane. n. 50 prevede un contributo a favore degli enti di area vasta per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di edilizia scolastica complessivamente di 470 milioni per il 2017, di cui 220 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane. Molte sono le deroghe davvero eccezionali previste alla disciplina contabile proprio per cercare di agevolare le Province che si trovano in una fase per così dire ancora transitoria, tra un percorso che era stato avviato con il con il compimento della riforma costituzionale che avrebbe visto la soppressione di questi enti ed il percorso attuale in cui invece si ridà pieno titolo a questi enti. le deroghe alla disciplina contabile, come anche la predisposizione del bilancio per la sola annualità 2017 e si spera che sia davvero solo per il 2017, perché le Province hanno bisogno di ritornare a programmare nel lungo periodo. Possono applicare per il 2017 l'avanzo libero destinato nel bilancio di previsione, c'è un'estensione al 2017 dell'applicazione ai bilanci di previsione delle quote di avanzo di amministrazione risultati dai trasferimenti da parte della Regione una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse. Alla Camera, oltre al testo base che già questo prevedeva, sono state inserite ulteriori misure: le Province e le Città metropolitane possono utilizzare i proventi delle sanzioni per la violazione del codice della strada ad esempio, gli oneri relativi alle funzioni di viabilità e polizia locale e per migliorare la sicurezza stradale. Per Per quanto attiene l'approvazione del rendiconto della gestione del 2017 si prolunga fino a cinquanta giorni il termine entro il quale l'organo regionale di controllo assegna al consiglio comunale e provinciale l'incarico all'approvazione al fine di evitare lo scioglimento dell'ente inadempiente. Sono stati dati anche ulteriori contributi; per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, l'articolo 20 prevede un contributo finalizzato all'esercizio delle funzioni fondamentali rideterminato in 180 milioni per le Province, 12 milioni per le Città metropolitane, un contributo straordinario per le strade provinciali di 170 milioni (all'inizio il contributo era previsto di 100 milioni) e tanti altri provvedimenti. Da quanto detto, si evince l'attenzione che è stata prestata alla situazione complessa in cui si trovano Province e Città metropolitane. Dal punto di vista del finanziamento, forse, si è fatto tutto il possibile, tenendo conto che questa è una manovra che doveva affrontare altri problemi di equilibrio. Forse però non è ancora abbastanza, se il presidente dell'UPI, in occasione della Festa della Repubblica, ha scritto una lettera al presidente Mattarella diceva che la legge di conversione del decreto-legge n. 50 rappresentava un'occasione importante, ma con amarezza constatiamo che il testo approvato alla Camera dei deputati prevede l'assegnazione di risorse insufficienti. Se il testo venisse approvato definitivamente in identica versione anche al Senato, in diverse Province dal Nord al Sud del Paese saranno inesorabili le decisioni di chiusure di scuole e strade, per l'impossibilità di intervenire per la messa in sicurezza. L'appello a intervenire non può però essere raccolto dal Senato, in quanto tra oggi e domani verrà posta la fiducia sul provvedimento. Si capiscono le esigenze di convertire velocemente il decreto-legge, ma non possiamo non rilevare, come peraltro ha già fatto il Presidente della Commissione bilancio, che il Senato ha votato la fiducia sulla legge di bilancio 24 aprile 2017, n. 50, quindi sono mesi che non può intervenire in alcun modo sulle norme che riguardano gli enti locali. Ciononostante uno spazio di intervento in Commissione è stato ritagliato e di questo ringrazio il vice ministro Morando che segue sempre con molta attenzione i lavori della Commissione e ha preso impegni per il Governo, esprimendo parere favorevole su ordini del giorno importante come il G/2853/61/5, a mia che impegna il Governo a prevedere nei prossimi provvedimenti utili o in sede di sessione di bilancio, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'adozione di misure finalizzate ad integrare le risorse finanziarie e di personale necessarie alle Province per esercitare le funzioni fondamentali previste dalla Costituzione e per garantire i livelli essenziali dei servizi di competenza dei rispettivi territori.

onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2853, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50, recante disposizioni recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione sulla fiducia, che avrà luogo questa sera, è stata ripartita un'ora e cinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo a partire dalle ore 9,30 di domani. Seguirà quindi la chiama, intorno alle ore 11. Dopo la votazione sulla questione di fiducia, l'Assemblea passerà alla deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73, in materia di prevenzione vaccinale, chiesta dal prescritto numero di senatori del Movimento 5 Stelle. Seguirà, come previsto dal calendario dei lavori, l'incardinamento del disegno di legge sulla cittadinanza con la sola relazione del Presidente della 1ª Commissione permanente sullo stato dei lavori. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno avranno luogo nella seduta antimeridiana di mercoledì 21 giugno, con inizio alle ore 9,30. Infine, il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame del disegno di legge di ratifica degli accordi di partenariato strategico, economico e commerciale tra l'Unione europea e il Canada, ove concluso dalla Commissione. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo davanti all'ennesima fiducia posta dal Governo Gentiloni Silveri, in continuità con le tante, troppe fiducie poste dal Governo Renzi, tanto da essere diventata un'arrogante prassi consolidata. Il decreto-legge è costituito da 67 articoli completamente eterogenei. Si passa dal trasporto agli enti territoriali, dalla finanza pubblica a quella locale. Si passa dal credito al lavoro, dallo sport (con il golf) e dal gioco d'azzardo alle ulteriori misure per il terremoto del Centro Italia, dove si registra un pauroso ritardo, con le macerie ancora da rimuovere e le casette assegnate con sorteggio. Fa specie che il relatore e alcuni colleghi della maggioranza abbiano parlato del provvedimento in toni trionfalistici, di manovra complessa e importante a cui è affidato il compito di sviluppare la crescita del Paese. Non ci saremmo dovuti trovare in questa situazione, anche perché, quando c'è una manovra correttiva, ci sono soprattutto tagli e un inasprimento della pressione fiscale, perché è evidente che i soldi da qualche parte si devono trovare. E i cittadini devono sapere che variamo questa manovrina obbligati dall'Unione europea, ma anche per il fatto che la legge di bilancio per il 2017, dal chiaro profilo elettorale-referendario voluto da Renzi, si scostava nettamente dagli obiettivi di indebitamento di medio termine. Renzi, insomma, ha cercato di finanziare le misure *pro domo sua* e del Partito Democratico, scaricando tutto sul debito pubblico, peraltro fallendo clamorosamente, come è successo per quasi tutte le riforme che ha varato: la legge Delrio, la buona scuola, il decreto salva banche, l'Italicum e in ultimo, per l'appunto, la riforma costituzionale. L'entità della manovra è pari allo 0,2 per che - come abbiamo letto - sono rappresentati da ben 2,8 miliardi di euro di maggiori entrate e da 0,3 miliardi di euro di tagli alle spese. Si vanno a recuperare i soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese, dunque l'economia reale e la gravissima situazione economico-sociale, che oramai nel Paese vige da troppo tempo. Lo fate tagliando i servizi ed estendendo lo *split payment*, creando ulteriori problemi di liquidità alle imprese che lavorano per la pubblica amministrazione e che stanno ancora aspettando i pagamenti promessi da Renzi. Lo fate tagliando gli investimenti; lo fate con ulteriori tagli agli enti locali; lo fate aumentando le accise sui tabacchi e sul prelievo erariale unico sui giochi, di cui peraltro diminuite il *pay out*, ovvero la percentuale di vincita. Lo fate in tanti altri modi, sino ad arrivare alla cifra di 3 miliardi e 100 milioni di euro richiesta dall'Europa. In questo contesto è grave che il Governo abbia comunque trovato 15 milioni di euro per superare criticità igienico-sanitarie e sanare insediamenti illegali di stranieri residenti sul nostro territorio, molto probabilmente campi *rom*. una grave discriminazione nei confronti delle centinaia di migliaia di famiglie italiane che, non per loro colpa, abitano in quartieri dove mancano totalmente fogne o qualsiasi opera infrastrutturale e di urbanizzazione per rendere degna la propria abitazione. Anche in questo caso emblematico avete confermato la vostra politica, che è tutt'altro che basata su rigore e legalità. In questo Paese, conosciuto negativamente al mondo per la sua tolleranza e per il buonismo imperante, possono starci comodamente i delinquenti, gli irregolari, gli immigrati clandestini e le cose irregolari, tanto arrivate voi a sanare tutto. Altro che rimpatri! Una protezione umanitaria non la negate quasi mai,

delle Province, con la quale avete non solo privato del voto i cittadini, ma soprattutto ridotto in povertà questi enti e dunque annullato i servizi sul territorio, date quest'anno 110 milioni di euro alle Province per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

È interessante poi sapere dove prendete parte di questi soldi: dal taglio alle Regioni delle risorse per il trasporto pubblico locale. È una vergogna. Lo ripeto ancora: andate dicendo che con questa manovra si rilancerà l'economia. Per favore: non prendete in giro gli italiani! Di fatto, il debito pubblico continua a salire. E lo segnalo dal febbraio 2014: da quando si è insediato il Governo Renzi ad oggi, ad oggi, esso è salito di 150 miliardi. Di fatto, la pressione fiscale continua a rimanere alle stelle. Di fatto, con questa manovra non ridurrete il numero di cittadini in povertà assoluta, che oggi tocca quasi 7,2 milioni di persone. Di fatto, con questa manovra non invertirete il drammatico *trend* del tasso di denatalità (il più basso d'Europa). Di fatto, con questa manovra, soffocando l'autonomia, limitate gli enti locali, impedendo di fare investimenti anche a quei Comuni virtuosi che godono dell'avanzo di bilancio, e quindi impedite di promuovere sui territori la crescita. È inutile che Gentiloni Silveri si lanci nello spazio dopo le correzioni in rialzo del PIL fatte dal Fondo monetario internazionale. Diciamo agli italiani le cose come stanno: in una congiuntura economica favorevole, l'Italia è terz'ultima per crescita tra i ventotto Paesi dell'Unione europea. E poi - cosa gravissima che sta mantenendo in apprensione le imprese - non disinnescate le clausole di salvaguardia firmate dal Partito Democratico, che dal prossimo 1° gennaio, se non si troveranno 15 miliardi, faranno aumentare l'IVA e le accise sui carburanti. Rinviate ancora tutto non avendo più un euro, perché avete sostanzialmente svuotato qualsiasi fondo del bilancio dello Stato. Sui *voucher*: avete sfruttato la manovrina anche per porre rimedio al pasticcio dei *voucher* che avete eliminato con decreto-legge, per evitare il *referendum* e dunque evitare di prendere un altro schiaffone dagli italiani, come quello che avete preso lo scorso 4 dicembre, quando è stata bocciata la pessima riforma costituzionale. Dimostrando di essere politicanti, avete però assunto una decisione irresponsabile, lasciando dalla sera alla mattina famiglie, piccole e medie imprese totalmente allo sbando rispetto a una programmazione - la loro - che avevano fatto. E avete pure lasciato i lavoratori occasionali senza guadagno. La reintroduzione dei nuovi *voucher* va sicuramente incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle famiglie, e come Lega l'abbiamo sostenuta, ma l'avete fatta male. La misura è insufficiente, come al solito: ne date la possibilità di utilizzo a pochissimi, certificando la totale inaffidabilità di un Governo e di una maggioranza che, ancora una volta, pensano di poter risolvere con un decreto-legge di mancette di mancette le reali esigenze del nostro Paese, peraltro innescando un problema politico al vostro interno. Vedremo se MDP voterà la fiducia oppure si assenterà, dovendo digerire i *voucher* dopo aver minacciato degli sfracelli. Mi avvio alle conclusioni dicendo che avete imposto nuovi tagli e sacrifici al Paese. Eppure, 3,1 miliardi - lo sottolineo - rappresentano i due terzi dei costi che sosteniamo per gestire in modo pessimo, scellerato e sciagurato l'immigrazione, in gran parte clandestina. Quest'anno spendiamo 4,7 miliardi: non lo diciamo noi della Lega, lo dice il ministro Padoan. Era qui che bisognava risparmiare, facendo cessare il *business*, troppo spesso illegale, dell'accoglienza. È una follia spendere 4,7 miliardi

che non scappano da guerre e persecuzioni, e li manteniamo per un tempo medio che supera i due anni. L'immigrazione è totalmente fuori controllo. E non solo non rintracciate e non rimpatriate gli irregolari, lasciandoli scorrazzare nel territorio italiano in preda alla criminalità e a fenomeni comprovati di radicalizzazione. Ma addirittura, vista la continua saturazione dei centri di accoglienza straordinari e dei centri SPRAR, che stanno proliferando ma con enormi problemi sociali e di sicurezza, da un po' di tempo a questa parte il Ministero dell'interno

Questa è una follia. Questa è una vergogna. Rispetto a questa politica totalmente inadeguata alle necessità dei cittadini, diremo "no" al provvedimento. I cittadini meritano di essere governati, e subito, da ben altre forze politiche, che hanno sicuramente molto più a cuore l'interesse comune degli italiani e non l'interesse del mondo intero, delle *lobby*, dei poteri forti, della propria poltrona, del proprio potere personale o di quello del partito (leggasi il Partito Democratico). È per questo che - come si augurano gli italiani - dobbiamo andare presto al voto, in modo tale che i cittadini possano scegliere finalmente, dopo troppi anni, il proprio Governo.

con le politiche di risanamento dei conti pubblici, particolarmente complesse e difficili anche in ragione di una crescita ancora troppo debole. Il Governo, prima Renzi e poi Gentiloni Silveri, ha agito bene, ma resta ancora molto da fare. L'Italia, anche e soprattutto per l'enorme debito pubblico, resta l'osservato speciale in Europa. Condividiamo la linea del ministro Padoan e del vice ministro Morando che hanno ottenuto con un paziente lavoro e senza fare inutili polemiche con le istituzioni europee - risultati importanti, riducendo la percezione di rischio nei confronti dell'Italia sia in sede europea che sui mercati finanziari, ottenendo ottenendo molte significative aperture anche in ordine alle clausole di flessibilità. Con questa manovra vengono parzialmente sterilizzate le clausole di salvaguardia, e ciò renderà più facile disinnescare l'aumento IVA con la legge di bilancio 2018. Al contempo, si è evitato di introdurre misure che potessero rappresentare una inversione di tendenza delle misure di risanamento. In considerazione della situazione difficile in cui si trova l'Italia, questo - a nostro parere - non è un risultato da poco! Gruppo per le Autonomie abbiamo attribuito assoluta priorità all'individuazione, nella manovra correttiva di finanza pubblica, di una rinnovata disciplina per la retribuzione del lavoro occasionale e per le famiglie. Come è noto, non abbiamo condiviso il carattere ideologico del *referendum* che ha portato all'obbligata soppressione dei vecchi *voucher*. La fase transitoria che ne è seguita ha determinato profonde incertezze e maggiori, non minori, penalizzazioni sia per le imprese e le famiglie che per i prestatori di lavoro occasionale. La normativa ora introdotta in sede di conversione non ripristina, purtroppo, la precedente disciplina dei *voucher*. Nel decreto-legge si è fatto però un primo passo inserendo norme che - a nostro giudizio - migliorano la situazione per le forme di lavoro che richiedono particolare flessibilità e che non possono coesistere con il vuoto legislativo che si era creato. Il contratto di prestazione occasionale rappresenta per le micro imprese, fino a cinque dipendenti, uno strumento adeguato e semplificato. E analoghe considerazioni debbono valere per l'introduzione del libretto telematico prefinanziato a disposizione delle famiglie in ordine ad asili nido, *baby sitting* e alla retribuzione di attività di assistenza o, su altro versante, a quelle senza fini di lucro, gestite dai privati. Riteniamo questo un primo passo, non ancora soddisfacente per non ancora soddisfacente per le ONLUS e per il sistema imprese. L'esame da parte della Commissione bilancio del Senato ha confermato altri aspetti certamente importanti per le nostre autonomie, come l'esclusione dello *split payment* per gli enti pubblici che siano gestori di demanio collettivo o beni di uso civico, la regolamentazione dell'affitto di alloggi da parte dei privati (il cosiddetto sistema Airbnb) e l'esclusione delle Province autonome dai bacini di mobilità per

e al conseguente aggiustamento contabile, sarà infine possibile dare finalmente il via alla costruzione del carcere di Bolzano, bloccato ormai da due anni per un intoppo burocratico, fermo restando che questa infrastruttura statale verrà finanziata con

Presidente, ho già argomentato sul tema in esame oggi, ma il tempo era tiranno. Colgo pertanto l'occasione per ribadire i concetti. Chissà mai che possano entrare più facilmente nelle coscienze.

due diversi modi di succhiare soldi agli italiani. Sia chiaro a tutti che il Movimento 5 Stelle chiede a gran voce più sicurezza sulle strade. Più sicurezza e meno multe è una cosa possibile ed è un principio contenuto anche nella normativa che ha introdotto gli autovelox. Gli autovelox, i *tutor* e i rilevatori ai semafori sono ammessi solo per finalità di prevenzione.

contrario, tutti corrono e l'unico risultato è che le istituzioni fanno cassa, perché la multa scatta, mentre la sicurezza peggiora

e dei trasporti ho chiesto l'apertura di un tavolo tecnico anche per verificare, tra le altre cose, le corrette procedure di omologazione di questi apparecchi, perché qualcosa non torna. Non ho però avuto risposta. Perché? Che paura ha di confrontarsi? riguarda i rilevatori ai semafori, i cosiddetti T-Red. Studi internazionali ci dicono che, per avere la massima riduzione degli incidenti, la luce gialla dovrebbe restare accesa otto, nove secondi. per cinque, quattro o tre secondi, la conseguenza sarà una diminuzione della sicurezza e un aumento delle multe - è esattamente quello che accade - perché un tempo limitato favorisce gli errori dei cittadini.

Servirebbe almeno un dispositivo che segnala quanti secondi mancano in quel preciso momento all'accensione della luce rossa. Ebbene, quel dispositivo esiste ed è il cosiddetto *countdown*, cioè il conto alla rovescia. Tale dispositivo non commina multe, ma - anzi - ti aiuta a evitare errori e rischi di incidenti

costano anche molto meno dei T-Red. Perché allora i Comuni non installano questi dispositivi? Abbiamo chiesto al Comune di Padova di installarli, almeno in aggiunta ai T-Red. La possibilità di multa rimane - non vogliamo proteggere gli scorretti - ma almeno viene ridotta.

Vi faccio un esempio: il Comune di Padova infligge agli automobilisti 10 milioni di euro in multe ogni anno. In Italia, nel 2016, le multe sono state in totale 1,7 miliardi. Il fatturato di questo *business* - per così dire - è aumentato dell'8,3 per cento nel 2016 e gli introiti sono aumentati del 45,6 per cento Forse gli italiani sono diventati tutti scriteriati? Sembra di no. Ad esempio, le multe per uso del telefonino sono diminuite, come quelle per guida in stato di ebbrezza. E perché nessuno faccia sciacallaggio, preciso che sono informazioni fornite dalla stampa vicina al PD. Il decreto legislativo n. 285 del n. 285 del 1992 stabilisce che la metà dei proventi derivanti dalle multe debba essere destinata ad interventi per la sicurezza: messa a norma delle barriere, *guard rail* salva motociclisti, automezzi per le forze di polizia, educazione stradale, segnaletica, i *countdown*. I soldi ci sarebbero, se lo scopo fosse davvero quello di salvare vite, ma è davvero questo ciò che il Governo vuole? Vuole aumentare la sicurezza dei cittadini o dare agli enti locali uno strumento per fare cassa e compensare i continui tagli nei trasferimenti? Lo capiamo in questa manovra ipocrita, perché nel decreto-legge è stato inserito da una manina l'articolo 4-*bis* che libera la destinazione d'uso dei soldi rastrellati con le multe, che saranno quindi facilmente di più: i Comuni sono incentivati a riempire di occhi elettronici strade e incroci. Su questo settore si buttano i fornitori delle apparecchiature e ovviamente alcuni enti locali spregiudicati, perché con 1,7 miliardi l'anno il piatto è ricco. Poveri siamo noi. Altra questione è quella dell'azzardo. Il Governo tenta in ogni modo di convincerci che è contro l'azzardo, ma in questa legislatura

e vedete anche voi che ci sono bar con sette-otto macchinette e non tutte sono occupate. E infatti il decreto-legge prevede che si vadano a togliere dove sono troppo affollate o rendono meno e non lo dico io, ma c'è scritto: «in relazione alla distribuzione regionale, sulla base della redditività degli apparecchi».

con puntate fino a 10 euro in pochi secondi. Ce ne sono 50.000 circa e in proporzione ottengono una raccolta sette volte maggiore delle sorelle da bar. Il Governo per queste macchine vampiro non prevede alcuna limitazione nella manovrina. Si tagliano i rami secchi da un settore saturo e si lascia prosperare quello che pompa maggiormente. L'aumento della tassazione che viene richiamato è fumo negli occhi, perché il Governo si prepara a mettere la museruola alle regole comunali

Emendamenti non ne hanno fatto passare uno che sia uno e si sa perché: è stata posta la fiducia. Allora ho presentato un ordine del giorno

oppure si stanno spingendo gli italiani da un mercato all'altro, da macchinette impattanti a macchinette ancora più pericolose, e cioè dalla padella alla brace. è poi la pillolina finale: oggi la normativa obbliga chi ha una sala bingo a rimanere nella sede espressamente indicata nella convenzione di concessione. Non può cambiarla a piacere:

in Romagna. Cercando su Internet si scopre che si troverebbe a Cesenatico e che l'emendamento è stato proposto da un parlamentare locale. Sarebbe gravissimo, signora Presidente, perché si tratterebbe di una norma *ad personam*. L'emendamento prevede di dare l'autorizzazione al trasferimento quando cause di forza maggiore rendono impossibile rimanere in quella sede. Tuttavia, se anche fosse, perché si dovrebbe cambiare la legge? Forse un imprenditore onesto, poniamo un barista, che ha la licenza ma gli scade l'affitto dei locali, trova chi può fargli una legge su misura? Qualcuno sostiene che, essendo diretti concessionari dello Stato, i titolari di sale bingo hanno diritto a maggiori tutele. sbagliato. Essere concessionari dello Stato comporta diritti e doveri e, tra i doveri, c'è il vincolo sulla sede, espressamente richiamato nella convenzione di concessione. Nessuno li ha obbligati a sottoscrivere quel patto. Se sono intervenute

richieste al Governo su questioni che mi sembrano molto rilevanti. ci sono articoli riguardanti i Comuni. La situazione degli enti locali in questo Paese è diventata davvero drammatica i Comuni, dai più piccoli a quelli medi, hanno subito tagli di oltre i due terzi dei trasferimenti. Non mi sento di condividere nella maniera più assoluta le scelte fatte dal Governo, perché - da un lato - si effettuano tagli alla generalità degli enti locali, mentre - dall'altro - le risorse risultanti dalle decurtazioni vengono assegnate in maniera clientelare. in particolare a dei provvedimenti che sono stati molto sbandierati, come quello sulla riqualificazione, che hanno assegnato 3,9 miliardi a progetti di riqualificazione delle periferie

certamente non imputabile all'amministrazione attuale, ma in generale alle varie amministrazioni che si sono succedute alla guida della città.

per esempio, alle Province che non fanno la manutenzione alle scuole; non vengono pulite le scarpate delle strade, gli asfalti sono tutti bucherellati come se ci fosse stata una guerra

Un'altra cosa che mi ha fatto ridere è la previsione della possibilità di procedere ad assunzioni attraverso la sponsorizzazione. Siamo veramente al ridicolo. Quante aziende oggi possono sponsorizzare le assunzioni di personale degli enti locali?

mancava prevedere che le aziende possono sponsorizzare le assunzioni agli enti locali. Deve provvedere lo Stato e, se non può farlo, cerchi di sprecare meno soldi. Infine, non posso non ritornare al discorso del terremoto.

la risposta non possono essere le magliette gialle. Non è cambiando il colore delle magliette da rosso a giallo che si risolvono i problemi di una zona fortemente danneggiata. I cittadini l'hanno vissuta come una presa in giro. Non è accettabile che un ex Presidente del Consiglio lanci idee di siffatto tipo. Per affrontare queste situazioni ci vuole senso di responsabilità. Bisogna capire cosa fare e oggi è difficile farlo, perché abbiamo avuto quattro decreti-legge emanati dal Governo. dal Governo. In discussione ci sono 13 articoli che riguardano le zone terremotate. Abbiamo avuto 8 decreti del capo della Protezione civile, accompagnati da 23 ordinanze.

a operare quando c'è una produzione di norme, leggi e Regolamenti che è alta 30 centimetri. Io, da sindaco, nell'ufficio tecnico ho un faldone in cui vengono raccolti tutti questi provvedimenti, ma è impossibile aggiornarsi. È peggio di un corso universitario, perché ogni giorno ne escono in quantità con i quali si modificano le scelte precedenti. Credo che un po' di confusione in questo senso sia stata fatta. C'è anche il discorso delle risorse. Non basta stanziare un miliardo di euro per procedere alla ricostruzione di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Poi, se la ricostruzione durerà tanto, chi volete che torni ad abitare in quelle realtà? Abbiamo "deportato" tutti i nuclei familiari colpiti dal terremoto e li abbiamo portati sulla costa. Ma se non c'è prospettiva di ritorno, la gente farà scelte diverse: comprerà appartamenti lì e iscriverà i propri figli alle scuole dei Comuni della costa. Qui vi assumete la grave responsabilità di distruggere mezzo Appennino,

delle scelte precise e puntuali in modo che la gente sappia a cosa ha diritto e cosa potrà avere nel termine. Il minimo bisogna metterlo lì. Si pensi a queste proroghe di termini di due mesi: è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale si possono fare i versamenti tributari senza sanzioni e interessi.

Risibili sono poi le risorse per la compensazione della perdita di gettito della TARI.

Questa misura, che prevede un indennizzo per le aziende locali se hanno subito una perdita del 25 per cento del fatturato nei quattro mesi successivi al terremoto, è una presa in giro, perché non comporta niente e non è di alcun aiuto a quelle popolazioni. Noi dobbiamo, invece, fare delle misure che consentano alle imprese che hanno un po' di buona volontà di insediare la propria azienda, di costruire uno stabilimento, di fare un investimento in quelle zone: altrimenti, quelle zone sono morte. Si poteva

ma quando ci sono argomenti importanti noi siamo sempre disponibili. Il presidente Berlusconi sul terremoto aveva detto: «Eccoci qua, siamo pronti, diteci cosa possiamo fare insieme». Il Governo, però, non ha voluto sentire ragioni e ora sta sbattendo il muso, perché quando un esponente del Governo va nelle Marche si trova di fronte una popolazione indignata, una popolazione che contesta tutto l'operato fatto dal Governo. Questa, quindi, è un'altra occasione persa.

il "tiro al bersaglio" atto a colpire i lavoratori e i delegati che erano in prima linea per la conquista dei diritti e della dignità del lavoro. Ci sono volute durissime lotte

Da alcuni anni questa pratica è tornata maledettamente di moda in Italia. Ormai non si contano più i lavoratori delegati che vengono licenziati con menzogne vergognose. E a venire licenziati sono sempre gli stessi. Pensate bene: chi pretende di tutelare i propri diritti e la dignità nei luoghi di lavoro. Praticamente, chi vuole difendere la democrazia di questo Paese.

e un compagno, un delegato che io conosco molto bene. È molto preparato ed è molto attento; un delegato che fa il proprio lavoro con passione, come ne sono rimasti purtroppo ormai pochi. Ed è forse proprio questo il motivo per cui anche questo delegato e questo compagno, cara Presidente, paga un prezzo così alto. Io vorrei dire a questo compagno di non preoccuparsi, perché la verità emerge sempre, e quindi di resistere, perché veramente viviamo un momento molto difficile. Questa politica, quella parte di politica che si riconosce ancora in questi valori, dovrebbe stare molto più attenta a questi temi, perché qui è in ballo - lo ripeto sempre - la democrazia di questo Paese. Quindi in bocca al lupo, Augustin, perché io credo che la verità verrà a galla, e resisti, perché c'è bisogno di resistenza, a partire dai luoghi di lavoro.

faccio seguito a una lettera che il sindaco di Valbondione ha già mandato al Ministro dell'interno lo scorso 27 maggio. Con tale

di 1.000 abitanti, è situato in un'area montana della Provincia di Bergamo ed è già in condizioni di forte svantaggio sotto l'aspetto di un'economia estremamente fragile, che ne ha caratterizzato gli ultimi decenni. Il prefetto ha comunicato al sindaco che verranno messe a disposizione da privati tre case vacanza, per un totale di circa 150 posti liberi. Questo mio intervento è proprio volto a significare come il *business* dei privati legato alla questione dei migranti sia arrivato anche in un paese dell'alta Val Seriana, con una totale mancanza di rispetto nei confronti dei residenti, che si trovano costretti a convivere quotidianamente con le problematiche generate dalla convivenza quotidiana. Dov'è l'impiccio, signora Presidente? Già dal giugno 2014 si sta vivendo una situazione di emergenza, tanto che attualmente nel Comune di Valbondione sono presenti 60 migranti nella piccola frazione di Lizzola, costituita da un nucleo di circa 200 abitanti, e altri 22 migranti nella frazione di Gavazzo, ove risiedono solo 31 persone. Quindi c'è uno sbilanciamento enorme nell'ambito di un sistema che ci vede assolutamente contrari, proprio come principio primo di attuazione di un sistema di accoglienza diffusa che è tale solamente sulla carta. Poi mi chiedo, signora Presidente, dove sia l'integrazione e se questi giovanotti, che

l'idea di aumentare la percentuale di atrazina nell'acqua per sistemare la questione della potabilità fosse applicata anche al caso dei migranti: appena si saranno superate le quote per ogni 1.000 abitanti, si modificherà la percentuale, in modo tale da poterne ancora nei Comuni. Quindi non credo ci sia una soluzione di sorta a questa problematica. Bene ha fatto il sindaco a scrivere ed è un problema che deve essere assolutamente collegato alla questione dello *ius soli*, che arriverà in questi giorni in Aula e su cui noi saremo sicuramente molto contrari.